L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

la quale preveda, accanto alla previsione della maggior rappresentatività a livello "nazionale", l'aggiunta della maggior rappresentatività a livello "territoriale",

a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. In assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali,

soltanto ricordare al Governo, nel momento in cui ci si accinge a dargli delega in tema di orario di lavoro, che la divisata soppressione della pausa di mensa di cui ci ha parlato il ministro Rotondi nei giorni scorsi costituirebbe violazione della disciplina comunitaria in materia, la quale impone che laddove la prestazione giornaliera superi le sei ore la pausa sia inderogabilmente

efficaci e proporzionate.

la gravità della sanzione deve essere rapportata al tipo di violazione ma anche alla dimensione, per cui la rendiamo proporzionata

stiamo leggendo l'articolo 1-*bis.* con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative», viene affrontato il caso dell'assenza di contrattazione nazionale regolatrice sul punto. In tale ipotesi, viene previsto che «In assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali, le deroghe possono essere stabilite nei contratti territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale».

con l'emendamento 5.202, è molto grave. Io e molti colleghi - non tutti perché la materia è controversa - siamo favorevoli alla flessibilità degli orari; non solo, ma siamo anche favorevoli a che la flessibilità degli orari sia regolata contrattualmente. Dico persino - e qui mi avventuro in un terreno delicato - che queste deroghe si possono fare anche a livello decentrato: giusto, Sottosegretario? Ma qui la cosa è veramente preoccupante! È la prima volta, che io anche se altri tentativi erano stati fatti - che questi contratti derogatori a livello aziendale possano essere fatti non solo, come sarebbe il caso, da sindacati collegati con le grandi le grandi centrali, ma anche da sindacati maggiormente rappresentativi su base territoriale. Il che significa che un piccolo sindacato rappresentativo nella provincia di Vercelli piuttosto che di Vibo Valentia - non ce l'ho con questi due centri può fare un contratto che modifica completamente l'orario di lavoro stabilito a livello nazionale. Trovo che questo sia devastante, e mi meraviglio del Governo, visto che abbiamo discusso molte volte della flessibilità e della derogabilità: derogabilità: l'ultima volta che ne abbiamo parlato mi sembra che il sottosegretario Viespoli fosse contrario; anzi, aveva fatto proprio una dichiarazione in tal senso. Quindi o è un equivoco che non ho ben compreso, oppure chiedo al Governo di chiarire

A questo punto, consentire la deroga ad un'organizzazione sindacale di qualsiasi entità, dimensione e genere significa eliminare sostanzialmente la disciplina della materia. modo si configura anche una violazione della direttiva comunitaria, che questo assolutamente non consente.

Il tema dell'orario in una azienda, in un contratto, in un settore, è un tema delicatissimo: ci sono regole, relazioni industriali che su questo punto possono mettere in crisi un'azienda, una società

ritrovarsi una maggioranza in grado di pesare sulla scena, si determina in un'azienda una situazione difficilissima, anche per la stessa azienda.

che destabilizzano l'organizzazione del lavoro, tutte improntate a un corporativismo che non risponde ad un'esigenza reale di rappresentanza e di organizzazione del lavoro. È questione, signor Sottosegretario, sulla quale davvero la invito a riflettere. Per questo, voto in dissenso dal mio Gruppo, rivolgendo una specie di appello: stiamo destabilizzando il sistema delle relazioni industriali. Non è una questioncella, quella in campo, attraverso l'orario si sta destabilizzando - ripeto - il sistema delle relazioni industriali. Credo sia gravissimo!

di questo provvedimento si rifletta su quanto è stato fatto adesso. Sono infatti convinto che c'è la massima disponibilità del Governo e del relatore ad interpretare un approccio di maggiore elasticità e maggiore possibilità di contrattazione. Si rischia però di rovesciare le carte. Se dovessimo avallare il principio secondo il quale una realtà

o non casualmente ma, comunque, per una serie di circostanze, rappresentano in modo maggioritario un gruppo di lavoratori. Sono convinto che né il Governo

in relazione alla confederalità della struttura dei meccanismi di regolazione delle relazioni industriali è cosa impossibile. Quindi, è una norma che favorisce, nella specificità

di dare soddisfazione al bisogno di finanziamento per i ricercatori. Il tema è sempre lo stesso: le risorse per i concorsi dei ricercatori sono già scarse in partenza. Con l'emendamento

Nell'università già da svariati anni non si fanno concorsi per i ricercatori e il rischio è che non vi sia nemmeno il minimo processo di riproduzione fisiologica. Se i ricercatori non possono fare i concorsi, l'università sostanzialmente sta ferma al palo.

molto assennata la scelta di sopprimere queste disposizioni per collocare l'intervento legislativo nella sua sede naturale, che è la riforma dell'università. Chiedo però che il Governo e i relatori adottino lo stesso criterio - più che ragionevole, dovuto - anche su altre materie. Tra poco ci troveremo ad affrontare una materia inerente al codice di procedura civile, che viene inserita in questo «minestrone» e non è stata neppure esaminata dalla Commissione giustizia. Spero che i relatori si rendano conto che la stessa ragione per cui un emendamento soppressivo in questa sede, al di là della valutazione dei contenuti della riforma processuale qui

Il tema è stato affrontato in quest'Aula anche in sede di discussione della finanziaria. Richiamo l'attenzione del Governo, che ha espresso un parere contrario, invitandolo a valutare l'opportunità di accogliere un ordine del giorno su questo argomento. La questione riguarda i posti di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori ex LSU (lavoratori socialmente utili) occupati prevalentemente per interventi di pulizia e mensa nelle scuole. Rispetto a questi lavoratori, che sono in carico a imprese di servizi vincitrici di appalti già nel 2003 e poi rinnovati nel 2006, non sono appostate nel bilancio dello Stato le risorse per la prosecuzione degli appalti per il 2010. Ricordo nuovamente che, in assenza di queste risorse, non solo circa 14.000 lavoratrici e lavoratori il 31 dicembre perderanno il lavoro (sono state avviate dal 1° ottobre le procedure di mobilità che scadranno il 31 dicembre), ma

le informazioni relative allo svolgimento del rapporto di lavoro siano rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non è chiaro come e perché, nella trasmissione dalla Commissione all'Aula, il termine "dalla" è stato trasformato in "alla", con il che si stravolge ovviamente l'intero significato della disposizione, cioè si annulla il principio di trasparenza totale. Poiché siamo tutti d'accordo che in Commissione abbiamo votato la preposizione "dalla", l'emendamento mira a ripristinare il testo dell'emendamento originario. PRESIDENTE. Invito il relatore

Signora Presidente, questo articolo, in sostanza, reintroduce la compartimentazione nelle carriere dei dirigenti pubblici. Ciò contrasta con un principio di buona amministrazione: innanzitutto, perché, se c'è un buon dirigente che proviene da una determinata amministrazione ed è utilmente destinabile ad un'altra, non c'è ragione di impedire, di scoraggiare, di disincentivare tale passaggio. Ma, soprattutto, ciò è in contrasto con tutta la logica della riforma delle amministrazioni pubbliche che il Parlamento ha varato pochi mesi fa.

mi stupisce che i relatori e il Governo si pongano contro se stessi, cioè contro quanto loro stessi hanno voluto in altra recente occasione. Non se ne comprende il motivo, se non per la soluzione di problemi,

sono, a loro volta, scorporati in due parti. L'intento di noi proponenti è quello di far ragionare anche sulla funzione del parlamentare.

anche sbrigativa, sommaria, vedremmo, caro Sottosegretario, che il sistema apicale di governo

che è un membro del Governo, che ha responsabilità complessive su tutto il settore e che, tutto sommato, risponde al popolo. riportare la sovranità popolare - che tanto si usa, ma a dismisura - ad essere elemento cardine della democrazia, non può essere che l'eletto, con un mandato di sovranità popolare, sia

Signora Presidente, preannuncio il voto favorevole del nostro Gruppo a questi due emendamenti, che affrontano un problema molto serio, quello del tetto alle retribuzioni dei manager pubblici - aggiungono i proponenti - delle società, in particolare delle banche, che ricevono sovvenzioni pubbliche in funzione di interventi anticrisi.

frettolosamente quella norma dal nostro ordinamento, ossia fecero una marcia indietro del tutto ingiustificata. Pertanto, l'approvazione dell'emendamento in esame consentirebbe di reintrodurre un principio, oltre che di contenimento della spesa - in una fase storica come questa

potendo interloquire in modo anche dubbioso su una parte dell'emendamento - in particolare l'ultima parte - che presenta qualche margine di opinabilità tecnico-giuridica,

gli emendamenti presentati dai colleghi Divina e Maraventano, intorno ai quali si è andata coagulando un'area di consenso molto vasta, toccano uno fra i problemi cruciali anche del più recente dibattito. Mi riferisco all'adeguatezza delle politiche retributive almeno per quegli enti e quelle compagnie che si trovino o investiti da significativi processi di riorganizzazione o che, essendo pubblici, dovrebbero ispirare a criteri di sana sobrietà repubblicana anche le loro politiche retributive. È di assoluta evidenza a chiunque di noi come si pongano, rispetto a queste proposte di intervento normativo, degli evidenti problemi di raccordo. Basti pensare alla straordinaria delicatezza di atti contrattuali stipulati tra una società e il suo *management* o i suoi amministratori, sui quali interverrebbe in maniera

di conversione dei loro emendamenti in ordine del giorno e - dall'altro - di rafforzamento del contenuto del medesimo ordine del giorno intercettando esattamente la direzione da loro così precisamente indicata.

l'erogante dovrà illustrare le ragioni di mercato che hanno condotto all'adozione della relativa politica retributiva. tutti i casi nei quali vi sia il superamento dell'obbligo di riferire al Parlamento, attraverso il Governo, delle ragioni di *compensation policy* che abbiano condotto ad un posizionamento del trattamento retributivo anomalo rispetto al parametro standard indicato dal Parlamento medesimo con questo ordine del giorno. Credo di poter sottoporre a tutti i colleghi una proposta che,

la sua proposta di trasformazione nell'ordine del giorno che lei ha testé letto - e che le chiedo di far pervenire alla Presidenza - riguarda

a rafforzare ulteriormente l'ordine del giorno. Si deve infatti individuare un percorso di confronto che arrivi poi ad una decisione, perché nessuno interpreti un'eventuale richiesta di ordine del giorno come un modo per non affrontare il problema, che c'è e che credo credo meriti un'attenzione, una puntualizzazione e un approfondimento rispetto all'impostazione normativa che emerge dagli emendamenti

Presidente, desidero rilevare che allorquando si affronta questa materia c'è sempre qualcuno che si incarica di suggerire una dilazione o una marcia indietro, non è la prima volta che questo avviene da parte dell'attuale maggioranza: i soli che ebbero il coraggio e la determinazione di affrontare il problema fummo noi, nei modi e nei tempi che tutti ricordiamo. con delusione della marcia indietro del senatore Divina, pur apprezzando gli argomenti che egli ha svolto. valorizzare la presa di posizione del senatore Divina e del relatore senatore Castro, che ha speso le parole che ha speso, credo sarebbe ragionevole conoscere, oltre che un testo preciso dell'ordine del giorno rafforzato, anche anche l'indicazione di un termine entro il quale il Governo - e mi rivolgo al sottosegretario Viespoli si impegna a riferire al Parlamento, magari nelle Commissioni competenti, quale sia la situazione delle retribuzioni dei manager pubblici, e non solo di quelli indicati nei due emendamenti, dato che a me risulta che anche in questa fase di grave crisi alcuni grandi boiardi hanno provveduto ad aumentarsi in modo consistente le retribuzioni,

Presidente, onorevoli colleghi, la questione posta dall'emendamento in esame e dal dibattito che ne segue è molto seria, anche perché noi, che facciamo parte del Parlamento, veniamo spesso additati, a torto o a ragione, come una casta beneficiaria di privilegi, con tutte le polemiche e le discussioni che ne conseguono, talvolta con fondamento, talaltra francamente senza, e viviamo in un mondo in cui molti manager

chi fruisce di finanziamenti pubblici deve avere un tetto che è il doppio della retribuzione parlamentare, per li rami si arriva a tutti: allora, anche l'amministratore del grande gruppo automobilistico tal dei tali, che deve trattare con la Merkel, con l'America e quant'altro, poiché l'azienda usufruirà certamente della cassa integrazione o di altri aiuti, dovrebbe essere trattato in un certo modo, il che poi farebbe sì che sul mercato non si troverebbero forse professionalità. Il tema merita attenzione, ci sono tetti che vanno posti, ma dobbiamo anche essere responsabili nell'immaginare che talune attività sia in società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, sia in società private aiutate dallo Stato richiedano un certo livello di professionalità. In quest'Aula,

giusta. Devo anche dire - e concludo - che recentemente di questi temi, e comunque delle retribuzioni di top manager - in quel caso, in una dimensione totalmente privata: pensiamo alle banche e alle crisi finanziarie perfino Sarkozy, la Merkel, i Capi di Stato e di Governo, e quindi anche il nostro Presidente del Consiglio, hanno discusso nei Vertici mondiali. Quindi, l'ordine del giorno sfiora questioni certamente serie. Leggere che prendono decine di milioni di euro o di dollari di liquidazione personaggi che hanno causato devastazioni finanziarie irrita tutti. Dopodiché, non facciamo confusione! Ci sono devastatori di bilanci pubblici e privati ma anche manager di elevate qualità

solo con emendamenti, ma con un ordine del giorno. Invito pertanto il Governo, nel contribuire alla stesura del testo, a consentire al Parlamento sistemi di monitoraggio. Non vogliamo fare demagogia ma garantire trasparenza. Ognuno deve essere davanti al Paese riconosciuto per le sue qualità, se ne ha, e per i suoi guadagni.

un ordine del giorno che, come è stato da ultimo indicato dal presentatore, e poi nell'intervento del presidente Gasparri, individui un percorso un richiamo alla responsabilità. Credo che ciò sia fondamentale, ed in fondo è questo il tratto distintivo del confronto che stiamo facendo:

c'è il tentativo di affrontare questioni estremamente delicate, che mettano insieme il merito, la professionalità, il senso di responsabilità, la sobrietà, il rigore e la ricerca di un punto di sintesi tra qualità e rigore che, soprattutto in questa fase, tutti responsabilmente siamo chiamati a dover affermare e fronteggiare. Con questo spirito il Governo è pronto a valutare l'ordine del giorno e ad assumersi anche la responsabilità del dopo ordine del giorno.

di acquistare strumenti informatici, dotati di apposita licenza, e di attribuire un credito d'imposta per i professionisti. Se i colleghi della maggioranza volessero sottoscrivere quest'emendamento per farlo diventare

di questo credito d'imposta è limitata sia nella sua attribuzione sia nella concorrenza finale, e potrebbe trovare facile accoglimento da parte dei colleghi che conoscono bene il mondo delle professioni e le necessità,

sarebbe anche opportuno, peraltro, estenderlo ad altre figure professionali e dirigenziali. Devo quindi esprimere un parere contrario.

forma anche una seconda casistica: non si può tornare indietro a seguito di contrattazione per un singolo individuo, perché magari è simpatico al dirigente o all'assessore, e non per gli altri che derivano da una contrattazione più collettiva. Quindi, l'articolo 11 è sbagliato. È un articolo che punisce soprattutto il lavoro femminile ed impedisce anche processi di ristrutturazione in settori che vanno ridotti. Chiediamo quindi

ricchi di concretezza del collega che mi ha preceduto devo aggiungere un altro tipo di motivazione, più relativa ad una dimensione di diritto.

della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Si dice che questa valutazione va effettuata nel rispetto dei princìpi di correttezza e buona fede: ora, la portata effettiva del riferimento ai princìpi generali non appare molto facilmente individuabile. sia pure con il limite riconosciuto della correttezza e della buona fede, questa disposizione consente di riesaminare, ed anche eventualmente di ritirare, provvedimenti emessi quando la trasformazione del rapporto di lavoro aveva la consistenza prima di un diritto soggettivo.

determina un accrescimento a favore della potestà della pubblica amministrazione a detrimento della libertà del dipendente.

sulle parole che mettiamo in fila e sulla ricaduta dell'approvazione di queste parole sulla vita delle persone. Non dovremmo mai dimenticare che relazione c'è tra le parole, le norme, gli emendamenti e la vita concreta delle persone. Stiamo chiedendo con questo emendamento di sopprimere

giustamente c'è anche un obiettivo dell'amministrazione di rispondere ai cittadini; ma, su un diritto già acquisito (si tratta, secondo me, di una norma illegittima), non è possibile intervenire nella vita delle persone, delle famiglie che si sono organizzate e delle donne che magari hanno deciso di crescere un figlio perché hanno una situazione familiare particolare, per dire «Tu, adesso, o torni a lavorare, o entri in difficoltà con l'azienda e con la struttura e magari puoi essere anche licenziato o messo in esubero». Credo sia una follia.

sconquassare vite personali e familiari, senza alcun giovamento. Signora Presidente, intervengo in dissenso dal Gruppo perché vorrei sottolineare la gravità di questo articolo, e annuncio che non parteciperò al voto.

di un'azienda o di una struttura pubblica. È sempre l'incontro tra queste due esigenze che determina una condizione lavorativa. Ora si

e di organizzare la propria vita in un certo modo, possa decidere all'improvviso, nel rispetto dei princìpi di correttezza e buona fede, che non significano assolutamente nulla,

La maggioranza in questo disegno di legge ha inserito proposte davvero incredibili, ma questa è tra le più incredibili. Per questa ragione non parteciperò al voto

colpita dalle argomentazioni che sono state sviluppate in Aula e che riguardano la gravità della ricaduta dell'approvazione di questa norma sulla vita di migliaia di donne italiane, vorrei chiedere l'accantonamento del voto su questa disposizione per una valutazione più meditata della questione che davvero - al di là delle esigenze

vi è stata la possibilità per chiunque abbia scelto il tempo parziale di organizzarsi in un certo modo (dal reperimento di un altro lavoro, all'assistenza di un ammalato, alla conduzione della famiglia)

conforme al relatore

1, prevede la possibilità per i dipendenti pubblici di essere collocati in aspettativa anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. si aggiunge che non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, Tutto ciò, dal nostro punto di vista, risulta in contrasto evidente con il dovere costituzionale del pubblico dipendente di servire la Nazione, di conformare la propria condotta e di ispirare le proprie decisioni e i propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico.

come potrebbe essere l'Agenzia delle entrate o l'ENAC, il quale chieda l'aspettativa e vada ad operare per un soggetto privato sottoposto ad indagine. In questa condizione e in questo lasso temporale egli potrà utilizzare le conoscenze acquisite nella pubblica amministrazione, compresi dati riservati relativi a quella stessa indagine, per costruire la difesa del nuovo cliente o datore di lavoro temporaneo. Ottenuto il risultato, potrebbe poi rientrare nella pubblica amministrazione. Questa situazione, che ho voluto rappresentare con un esempio, può essere immaginata in diversi campi della pubblica amministrazione. È per questo motivo che chiediamo la soppressione dell'articolo 13.

professionista che si pone in aspettativa può diventare concorrenziale nel suo lavoro esterno nei confronti della pubblica amministrazione? Vogliamo tutelare sia la sua libertà di mettersi in aspettativa, che gli interessi della pubblica amministrazione? Il mio intendimento

compattezza della maggioranza un impegno a rivedere il tema delle incompatibilità. Mi sembra una questione ragionevole.

Presidente, questa disciplina ha un percorso particolarmente lungo, che si ricollega si ricollega al Testo unico degli impiegati civili dello Stato n. 3 del 1957 e alle successive disposizioni. Il provvedimento di aspettativa non radica posizioni di diritto soggettivo, nel senso che il dipendente può semplicemente presentare l'istanza,

L'ulteriore provvedimento ministeriale definisce la collocazione in aspettativa. È del tutto evidente che, nell'adozione del provvedimento, l'amministrazione, indipendentemente da ciò che non è scritto in questa norma, deve valutare la salvaguardia dell'interesse pubblico e un eventuale conflitto degli interessi, perché è principio generale del diritto che la pubblica amministrazione sia organizzata su elementi di esclusività dell'azione amministrativa. Esprimo

sta nel fatto che l'impegno finale è una sorta - mi permetto di definirlo così - di emendamento mascherato che prosegue la critica alla legge in discussione. Quindi, mi sembra un ordine del giorno che in realtà non è tale. Ciò è legittimo dal punto di vista politico ma è altrettanto legittimo che il Governo affermi che, se davvero c'è l'obiettivo di costruire

mi chiede e mi propone una riformulazione, la voglio vedere e valutare. Credo, d'altra parte, sia interesse del Governo, oltre che dell'opposizione che è forza di governo si batte su questo, la tutela della pubblica amministrazione. Relatore Saltamartini, è stata eliminata la vecchia legge sulle incompatibilità, stata eliminata la vecchia legge sulle incompatibilità, e questo va bene, ma non è stato previsto niente altro. Quindi è inutile che lei parli della tutela della pubblica amministrazione, perché si sta facendo il contrario: non c'è alcun paletto. Vogliamo riformulare in modo un po'

nelle sue dichiarazioni di poc'anzi. C'è un'ambiguità, un non detto, un tentare di non affrontare la questione. Il punto è semplicissimo: si tratta di fissare un punto di principio, e bene fa la senatrice Incostante a chiedere la riformulazione. Voi cosa pensate? Qual è il punto sul quale articolate articolate e articolerete la vostra azione legislativa? Quello di abolire ogni incompatibilità e di presumere l'impossibilità che si produca un conflitto di interesse, ovvero quello di partire con una disciplina che azzera tutte le incompatibilità (che è un errore:

quello di respingere un ordine del giorno che ha un unico merito essenziale, ossia porre la questione? È possibile in questo Paese prevedere una disciplina che regoli incompatibilità e conflitti di interesse tra l'appartenenza alla pubblica amministrazione e l'esercizio di una libera professione? Questo è il tema Questo è il tema sul quale il Governo e la maggioranza si devono pronunciare. Possono anche assumersi in quest'Aula la responsabilità di dire che per loro, in radice, il principio da affermare è l'assoluta libertà e quindi l'assenza di ogni incompatibilità e conflitto di interessi. Quello che non è ammissibile è dare un colpo alla botte e un colpo al timpano, cioè lasciare nell'indeterminatezza e nell'ambiguità una questione così delicata della quale il Parlamento torna ad occuparsi dopo la riforma che era stata introdotta.

che non altera il sistema delle incompatibilità presenti nella struttura del rapporto di lavoro all'interno della pubblica amministrazione. Le incompatibilità rimangono per il settore del pubblico impiego privatizzato, già disciplinate dal decreto legislativo 30

dipendenti statali dell'aggregato complesso del pubblico impiego possano chiedere di essere collocati in aspettativa per un anno. Questa misura è a discrezione dell'amministrazione; la posizione giuridica dei dipendenti è di mero interesse legittimo.

quali attività di impresa o professionali i dipendenti pubblici collocati in aspettativa, quindi sottratti al rapporto di lavoro, possano esercitare. Quindi, si tratterebbe, secondo le tesi dell'opposizione, di introdurre in una norma che ha le caratteristiche *relatore*. Si tratterebbe di individuare all'interno di una fattispecie generale e astratta tutti quei casi umani che riguarderebbero lo scibile o la volontà dei dipendenti pubblici di svolgere attività professionali e imprenditoriali: è un'attività materialmente impossibile. Dopodiché, l'incompatibilità riemerge nell'ipotesi in cui il dipendente che è stato collocato in aspettativa, che ha svolto l'attività professionale e imprenditoriale, richieda di tornare al servizio della pubblica amministrazione. In quel caso l'incompatibilità avrebbe efficacia. La disposizione comunque non elimina le incompatibilità. Le amministrazioni dovranno garantire il corretto esercizio dei canoni costituzionali, che sono quelli dell'imparzialità, dell'efficienza, dell'esclusività della pubblica amministrazione. Intervenire su una norma costituzionale come quella dell'articolo 97 è un mero pleonasmo. Per questo, ribadisco il parere contrario su questo ordine del giorno, che potrebbe essere accolto

Quest'Aula ha più volte espresso un consenso unanime nei confronti della peculiarità del personale di cui ho parlato.

generoso, ad esempio, dei nostri Vigili del fuoco nelle ripetute circostanze di calamità naturali oppure nei confronti delle Forze di polizia a ordinamento civile o militare nella lotta contro la delinquenza e la criminalità o, infine, verso i nostri militari che operano in condizioni rischiose nei vari teatri operativi del mondo e in Italia a supporto delle Forze di polizia. Ma la specificità è anche altro. Infatti, questo personale è legato da obblighi che nascono da norme disciplinari che valgono soltanto per loro, svolge attività senza limitazioni di orario

Ebbene, questo emendamento che il Partito Democratico ha presentato vuole dare concretezza a questa specificità

aspettative e alle loro esigenze, ma soprattutto che è in armonia con quanto quest'Aula in più circostanze ha voluto riconoscere nei confronti delle Forze armate,

precisazione. Con l'articolo 14 del provvedimento si riconosce per la prima volta nella struttura della pubblica amministrazione, nel comparto sicurezza e difesa, cioè quanto al personale che ancora risulta legato ad un rapporto giuridico strutturato sulla base della legge, contrariamente alla alla delegificazione e alla natura privatistica e contrattuale del restante personale del pubblico impiego, questo criterio della specificità, in forza del quale le atipicità delle prestazioni lavorative, il rischio professionale (anche della vita) dei militari, delle forze dell'ordine e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, devono trovare un riconoscimento specifico livello contrattuale. La norma che introduciamo con l'articolo 14 prevede, senza fondi aggiuntivi, questo riconoscimento di *status*. Giustamente il senatore Del Vecchio e gli atti firmatari di questo emendamento prospettano l'esigenza di finanziare questa specificità. Tuttavia, in questa fase il provvedimento non può trovare un idoneo finanziamento proprio per le esigenze generali della finanza pubblica.

In seconda analisi, l'emendamento non è determinato, nel senso che la costituzione di questo fondo, da ripartire secondo specifici criteri dal Governo, andrebbe allocato nei livelli di contrattazione, che possono essere il livello nazionale, il livello della produttività di ogni singola amministrazione, addirittura attraverso l'accordo nazionale quadro.

di valutare l'impiego dei fondi relativi al rientro dei capitali all'estero con lo scudo fiscale, se una parte possa essere assegnata a finanziare il principio di specificità. In ordine all'emendamento 14.0.200, che è stato trasformato in ordine del giorno dalla senatrice Maraventano,

alla ricerca di una copertura finanziaria magari diversa rispetto a quella individuata nell'emendamento stesso. Con questo spirito chiedo al al presentatore, se lo ritiene, di ritirare l'emendamento, o almeno di trasformarlo in un ordine del giorno, che sarei pronto in questo caso ad accogliere fin da subito. ringrazio il signor Sottosegretario per le sue precisazioni. Non credo sia opportuno ritirare l'emendamento, e quindi

con l'espressione "a verificare la possibilità", che forse formalmente è più rappresentativa di quanto vogliamo dire. Con queste modifiche vorrei apporre la mia firma, se la collega acconsente, al

per il Gruppo del Popolo della Libertà l'articolo 14 è una parte molto importante di questo peraltro rilevante disegno di legge. Infatti, riconosciamo finalmente la specificità

possiamo sancire la specificità di coloro che, uomini e donne, in divisa, in Italia e all'estero, svolgono una funzione delicatissima per la nostra sicurezza. È ovvio che il riconoscimento della specificità non deve essere soltanto un fatto di ordine morale, ma una scelta ordinamentale che può poi giustificare scelte di natura economica e normativa, che siano adeguate alla specificità delle forze dell'ordine e del mondo militare. In questo senso, condividiamo anche lo spirito dell'ordine del giorno che recepisce un emendamento

all'insegna di un principio di specificità che da questa legge viene rafforzato, abbiamo già aggiunto 100 milioni di euro per il rinnovo contrattuale del personale del mondo della sicurezza e militare. Ci rendiamo conto che di risorse ne servono altre e ci auguriamo che nel prosieguo dell'esame della legge finanziaria, sia alla Camera che al Senato, se ne possano individuare. Al di là però del contratto o del riconoscimento momentaneo, con questa legge riconosciamo in maniera permanente la specificità delle forze dell'ordine e dei militari nell'ambito del mondo del lavoro. È una norma che viene introdotta per sempre nell'ordinamento e credo sia un atto

in tralice il senatore Gasparri - è chiaro che una norma come la specificità o si sostanzia di risorse oppure è in qualche modo soltanto un bel riconoscimento. La richiesta forte

esserci risorse essenziali: 100 milioni di euro, tra l'altro con coperture da verificare, sono una goccia rispetto ai tagli fatti sui bilanci delle forze dell'ordine.

sui trattamenti relativi al personale deceduto in attività di servizio istituzionale che è già stato operato dal decreto-legge sulle missioni internazionali in via di conversione da parte del Parlamento.

perché gli emendamenti che verranno esaminati nell'ambito del decreto per la prosecuzione delle missioni fuori area sono ancora all'esame della Commissione e, da quanto è dato sapere, qualcuno di essi potrebbe essere giudicato non ammissibile

che purtroppo siamo chiamati a vivere giornalmente con il personale militare che opera in determinate circostanze. Mi riferisco, ad esempio, alla strage di Nassiriya, che che originò situazioni veramente difficili per garantire la promozione a tutti coloro che purtroppo erano risultati vittime di quella strage, e mi riferisco

Questo emendamento consentiva a quel personale di poter rimanere in servizio e quindi dava un riscontro immediato alla loro dedizione e al loro impegno per il Paese.

come risulterà comprensibile ricorro a questa opportunità regolamentare parlando in dissenso dal Gruppo

che il relatore Saltamartini ha fornito dando risposta all'intervento del senatore Del Vecchio denuncia di fatto una attendibilità di quelle affermazioni.

dell'emendamento del senatore Del Vecchio potrebbe trovarsi già in altre norme di fatto si intende scientemente evitare di assumere un atteggiamento preciso. Pertanto oggi, nonostante la dichiarazione del relatore, come Senato stiamo dicendo no alla proposta di sanare questa vergogna: vergogna: è l'espressione più evidente dell'incoerenza tra ciò che il Governo afferma nei confronti dei militari e ciò che poi effettivamente fa. D'altro canto, anche la grande ipocrisia sulla specificità testimonia dell'indisponibilità del Governo a farsi carico di questi lavoratori della pubblica amministrazione. Ciò che dispiace - e non poco è che l'atteggiamento politico complessivo che informa questo disegno di legge è assolutamente individuabile come un atteggiamento ostile al lavoratore. In maniera esplicita ed evidente, spesso anche in maniera molto sottile ed artificiosa, si sta cercando di creare un contesto complessivo per limitare le libertà del lavoratore, contenere e comprimere le tutele che per molti anni il lavoratore ha avuto grazie a serie, importanti ed efficaci azioni sindacali

oggetto dell'articolo 15-*bis* sono le misure atte a garantire le pari opportunità, il benessere di chi lavora, in assenza di discriminazioni, nelle pubbliche amministrazioni. Il presente articolo modifica gli articoli e 57 del Testo unico sul pubblico impiego. In particolare, la lettera *c)* prevede l'unificazione, in un solo organismo, denominato Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, di tutti i comitati per le pari opportunità e paritetici sul fenomeno del *mobbing*. Se in linea di principio una semplificazione e un accorpamento degli organismi di controllo possono sembrare positivi, è tuttavia da notare che la disposizione in parola scavalca l'autonomia contrattuale. Inoltre, poiché riteniamo che la materia dovrebbe costituire oggetto di un disegno di legge organico, chiediamo che venga soppressa da questo provvedimento.

L'aspetto formale è stato testé illustrato dalla senatrice Carlino: c'è un superamento della contrattazione collettiva. L'aspetto sostanziale riguarda

i comitati paritetici sul *mobbing* svolgono una diversa funzione. Quindi, in questo momento storico non se ne giustifica l'accorpamento. Questo tanto più se si considera che proprio nello stesso disegno di legge in esame si prevede

attraverso l'abolizione dei comitati aboliamo anche la possibilità di un ricorso a un diritto antidiscriminatorio che chiaramente è violato con la norma sul *part-time*. Il diritto antidiscriminatorio non è un'opinione, perché ormai è radicato nel nostro ordinamento e costituisce un diritto costituzionale su cui non si può incidere. Inoltre, tutta questa materia organizzata in maniera così confusa finirà con aumentare la conflittualità in sede giurisdizionale,

il parere del relatore.

I comitati per le pari opportunità, le loro azioni, le loro esperienze e talvolta anche le loro significative prassi si annacqueranno in un unico comitato,

statuito tra le parti, con suoi compiti e funzioni, che non può essere confuso con altri comitati. Quindi, con questa legge arrechiamo un danno ai comitati per le pari opportunità

Tra l'altro, osservo come in molte amministrazioni pubbliche siano impigriti e rattrappiti sia il comitato antimobbing, sia il comitato per le pari opportunità. Tale scelta strategica trova riscontro non a caso nei migliori esempi internazionali, comitati antimobbing e, laddove si manifestano problemi di integrazione razziale, anche i comitati per l'integrazione, si fondono sulla piattaforma soda e solida della pari opportunità, nella quale si innesca la congiunzione della fase difensiva,

in modo da garantire che siano per vocazione in maggioranza i rappresentanti del genere femminile. Chiedo alle colleghe se accolgono la mia proposta. Almeno paritaria per il genere femminile:

il termine «almeno» assume un significato solo se il testo legislativo fa riferimento al genere femminile, ma in questo caso il testo fa riferimento a entrambi i generi. Quindi, l'introduzione

Presidente, le argomentazioni e le risposte del relatore su questo emendamento non ci hanno convinto. Anch'io vorrei rivolgermi, oltre che al Governo e al relatore stesso, alle donne

che so essere molto sensibili ai temi della parità e delle uguali opportunità. Forse stanno sottovalutando la questione. Non è solo un fatto burocratico. È un fatto sostanziale, come ha detto poc'anzi la senatrice Della Monica, ed è una soluzione che va oggettivamente a depotenziare organismi che sono nati per combattere le discriminazioni di genere. Sappiamo che nel nostro Paese le discriminazioni aumentano ogni giorno di più, non diminuiscono, a partire dalla disparità salariale anche nella pubblica amministrazione.

che cambia la composizione del Comitato nazionale per l'attuazione dei princìpi di parità, diminuendone l'autonomia e anche in questo caso l'efficacia, il risultato si traduce

una sfida nei confronti delle donne e delle loro aspirazioni ad una reale parità e a reali ed uguali opportunità.

le preoccupazioni suscitate dalla trasformazione in un organismo in cui le questioni della parità riferite al genere finiscono per essere una delle tante e possibili discriminazioni. Forse però è proprio questo il punto. La differenza di genere e i problemi ad essa collegati non sono una delle tante possibili discriminazioni: sono problemi che hanno a che vedere con la metà degli abitanti di questo pianeta, le cui discriminazioni vengono sottaciute e, se del caso, spacciate per una delle tante discriminazioni. Ci sono i portatori di handicap, gli stranieri, le donne. Non

l'opera di razionalizzazione alla base del nuovo articolo 15*-bis*, ritengo comunque che sia importante riaffermare la validità e il ruolo dei comitati per le pari opportunità nelle pubbliche amministrazioni,

far riflettere le colleghe dell'opposizione, che con passione e veemenza hanno posto il tema del *mainstreaming* delle pari opportunità

contrariamente a quanto sostenuto dalla senatrice Adamo, esso non inficia e soprattutto non indebolisce il tema delle pari opportunità; anzi, lo rafforza. Il tema del *mainstreaming* passa oggi modernamente attraverso le tante difficoltà e le tante pari opportunità che dobbiamo saper garantire nel momento in cui legiferiamo su una materia così delicata, non solo in riferimento alle relazioni industriali ma anche alla centralità del tema del lavoro

oltre all'arricchimento culturale di ciascuna di noi e di tanta parte di generazione femminile cresciuta all'interno di quel contesto, cos'altro pensiamo di aver di aver ricevuto da questo processo, che è finito per diventare nel tempo, anche in breve tempo, solo una modalità burocratica?

chiunque è in difficoltà, di chiunque resta indietro o rischia di restarlo. Penso sia più giusto guardare alle pari opportunità di oggi e non a quelle di 20 o 30 anni fa e che quindi questo strumento vada rafforzato ulteriormente allargando lo spettro; spettro; altrimenti il comitato per le pari opportunità continuerà ad essere quello che è già diventato, un gineceo riferito solo alle donne, dove solo le donne possono parlare tra loro.

sottolineare ai colleghi di quest'Aula come il testo proposto dal relatore possa essere largamente condivisibile. Lo dico anche dai banchi dell'opposizione, senza aver timore di farlo rispetto a ciò che sto asserendo. D'altra parte, l'Europa da tempo ha unificato nel discorso di pari opportunità anche la non discriminazione e ha svolto in questi anni un'azione forte e incisiva a livello culturale per assommare alla pari opportunità un contesto molto più ampio, che è quello appunto della non discriminazione, che va ben al di là delle battaglie della pari opportunità, che riguarda semplicemente il genere. C'è qualcosa di più che dobbiamo considerare: una cultura vasta della non discriminazione e della pari opportunità, che va ricondotta a sintesi e non spezzettata in una serie di comitati; però va ricondotta a sintesi non solo al livello di cui noi ci stiamo occupando, ma anche a livello politico generale. La pari opportunità e la non discriminazione anche nel nostro Paese richiedono un Ministero con portafoglio; richiedono una Commissione parlamentare. Se ne fanno tante e tanto inconcludenti, si dovrebbe fare una Commissione parlamentare per la pari opportunità e la non discriminazione che accolga e valuti tutti i temi che oggi devono garantire a tutti i cittadini un adeguato comportamento da parte della legge, da parte del Governo, una sicurezza di parità e di non discriminazione in tutti gli interventi legislativi che mettiamo in essere, una politica che incentivi la pari opportunità e la non discriminazione

rispetto assolutamente non solo l'esperienza, ma anche la passione a cui ha fatto riferimento il senatore Castro, relatore del provvedimento, sul tema delle pari opportunità e anche le esperienze pratiche e concrete alle quali, con la sua attenzione, ha dato vita. Mi lasci dire che, se la spiegazione del cuore di questo articolo sta nella razionalizzazione organizzativa della materia, qualche dubbio e qualche perplessità ce l'ho sulla coerenza di questa razionalità organizzativa. Non vorrei che nella stessa razionalità organizzativa stesse la giustificazione della revocabilità del *part-time* e soprattutto non capisco come il Governo, con il decreto legislativo n. in attuazione peraltro di una direttiva, abbia recentemente allargato e di molto rafforzato l'ufficio della consigliera di parità, cioè esattamente l'equivalente nazionale di quello che le commissioni opportunità sono all'interno della pubblica amministrazione, oltre che nell'impiego privato. Che senso ha agire da una parte allargando, e quindi radicando la specificità della commissione nazionale, e dall'altra andando

La questione è un'altra ed è squisitamente politica e direi - meglio - una questione squisitamente culturale. Ciascuna di noi, anche la collega Bonfrisco, che ovviamente deve fare il suo mestiere in quest'Aula, e le molte senatrici che sono qui, a cominciare da Ida Germontani, sanno bene che la questione, per quanto riguarda le politiche di pari opportunità, nel nostro Paese ha sempre rischiato di essere declinata soltanto come lotta contro la discriminazione e azione di tutela contro una debolezza, che è la debolezza femminile. Io credevo che, proprio adesso che sulla pubblica amministrazione e sulla sua modernizzazione questo Governo punta tanto, fosse riuscito a passare quel pezzo del messaggio che migliaia e migliaia di donne italiane testimoniano ogni giorno ovunque (nella scuola, nelle università, nelle professioni, nella pubblica amministrazione), per il quale il problema della pubblica amministrazione oggi non è quello di razionalizzare questi organismi e farne uno che si occupa di tutte le discriminazioni, di tutte le debolezze, di tutte le violenze, e tuteli le donne, i portatori di handicap, l'insieme dei soggetti che subiscono violenza (cosa sacrosanta), è quello di prendere atto, nella riorganizzazione della pubblica amministrazione, della partecipazione, sia pure ridotta e sia pure segnata dall'esclusione di genere, delle donne italiane e cercare di fare in modo che il potenziale che rappresentano diventi una delle molle essenziali della modernizzazione, della nuova capacità e della nuova abilità dell'amministrazione italiana. La norma così come è - lasciatemelo dire - prosegue nelle politiche di tutela rispetto alle quali siamo sempre in bilico. Insomma, tanto per essere chiari, sono coautrice, quindi orgogliosa, delle norme che sono state costruite in questo Paese sulla violenza sessuale, sui maltrattamenti, sul *mobbing*; però vorrei che - per una volta - ci rendessimo conto che qui non stiamo parlando di debolezze, ma, insieme, di forza. E se questa appare come un ingombro è perché è esattamente così. Deve essere un ingombro tale dobbiamo rappresentare con una tale vivezza la presenza delle donne nella pubblica amministrazione da non cercare la scappatoia che mortifica la possibilità di utilizzarle al meglio, per rendere più efficiente, più vicina ai cittadini, più moderna e più competente la pubblica amministrazione

non moderno, non interessante per il funzionamento della pubblica amministrazione e non qualificante per la riforma della pubblica amministrazione; è un approccio inconsapevole, timido, addirittura forse impaurito

cercando di comprendere come attraverso questa strada si riesce a dare nuovo impulso all'amministrazione pubblica, oppure rischiamo di fare una cosa che forse sarà in linea con quello che fa qualche altro Paese ma che, francamente, rispetto al giacimento che abbiamo di intelligenza, competenza, abilità, voglia di fare e determinazione, è riduttivo e assolutamente inadeguato al compito che abbiamo dinanzi.

Presidente, solo per ricordare brevemente che l'età pensionabile dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale ha già appassionato quest'Aula

l'età lavorativa reale a 40 anni di contributi effettivi, di servizio effettivo. Nel passaggio tra Senato e Camera ritornò quella finestra pensionabile completamente stravolta, tant'è che anche il ministro Brunetta ha tentato quest'anno di porvi rimedio. Il richiamo ai 70 anni qui formulato,

ad approvarlo nella formulazione che abbiamo descritto, ripensando all'originario momento di intesa di quest'Aula, che era sui 40 anni di servizio effettivo come limite dell'età pensionabile per i medici del Servizio sanitario nazionale.

Signor Presidente, l'emendamento 17.1 è volto a sopprimere l'articolo 17, che reca una delega al Governo ai fini del riordino della disciplina in materia di congedi, aspettative e permessi spettanti ai lavoratori dipendenti pubblici e privati. Si segnala che questo articolo si abbatte come una scure in modo indiscriminato non solo su coloro che possono aver abusato delle norme, ma anche su coloro che ne usufruiscono in maniera pulita, limpida e corretta. Sulla lotta ai falsi invalidi, su cui naturalmente non si può non essere totalmente d'accordo, faccio presente che l'articolo 80 del decreto‑legge n. 112 del 2008 prevede un piano di 200.000 accertamenti di verifica da cui dovrebbero addirittura derivare 100 milioni per i prossimi tre anni. Quindi, chiediamo che si applichi tale piano per l'accertamento piuttosto che modificare la legge.

considerato negoziale - quello della ridefinizione, laddove è ritenuta necessaria, dei modi di accesso ad una serie di diritti che sono il presupposto del godimento dei permessi a cui la delega accenna genericamente - venga nuovamente trasformato in ambito normativo, peraltro peraltro già disciplinato in maniera precisa e puntuale, i cui contenuti recuperano la storia di un percorso di lotte per l'affermazione di diritti soggettivi, in particolare di diritti delle donne e delle persone con difficoltà. Quindi, crediamo che l'intento - anche in questo caso affermato come intento di riorganizzazione, di maggiore efficienza - posto alla base della motivazione della delega sia in realtà

la pubblica amministrazione, così come i datori di lavoro privati abbiano tutti gli elementi e dispongano di tutti gli strumenti necessari per contrastare gli abusi che, ovviamente, ledono l'impianto dei diritti. Ricordo a titolo di esempio la campagna promossa qualche tempo fa dal ministro Brunetta contro i permessi concessi ai donatori di sangue. Ora, se il tema è l'abuso di alcune categorie di permessi, non è necessario, anzi è profondamente profondamente controproducente rivedere tutta la disciplina. Al contrario, occorre che la pubblica amministrazione e gli organi di controllo anche in ambito privato - quindi l'INPS - mettano in atto

la ridefinizione nell'ambito di una delega amplissima dei presupposti oggettivi e soggettivi che stanno alla base dell'accesso a queste tutele esponga

la necessità di non aprire un conflitto sociale, e la necessità di non riaprire un contenzioso su una materia già regolarmente disciplinata dalle leggi. Un'ultima sollecitazione è contenuta nell'emendamento 17.3: almeno si sottraggano sottraggano all'ambito della delega, per rimetterli completamente alla contrattazione collettiva, i permessi relativi a motivi familiari. In quest'Aula più volte il ministro Sacconi ha avuto modo di richiamare il fatto che le famiglie attraverso la gestione dei permessi

L'articolo che stiamo esaminando intende delegare al Governo un riordino della materia e, più precisamente, il coordinamento formale e sostanziale,

riordino della normativa sui permessi. Questa materia non è oggi sparpagliata in una pluralità di interventi legislativi, come tanta altra parte della materia del diritto del lavoro, ma è già oggetto di un Testo unico, unico, il decreto‑legislativo n. 151 del 2001, che ha esattamente coordinato e riordinato

grande problema che dobbiamo porci a questo riguardo, poi, è che tutti questi permessi e congedi, che svolgono una funzione di grande rilievo sociale, sono disegnati di un modello di rapporto di lavoro che è quello del pubblico impiego e della grande impresa. Il problema è rendere accessibili

che siano davvero godibili anche dal dipendente dell'azienda con cinque dipendenti, dal dipendente della bottega.

Presidente, sull'articolo 17 mette conto di sottolineare la portata e la *ratio* *legis* della normativa che viene proprio perché si tende a ridefinire i presupposti oggettivi e soggettivi dei congedi e dei permessi per avvicinare il rapporto di lavoro pubblico a quello di lavoro privato. La materia riguarda quindi non solo il settore pubblico, ma anche quello privato. Peraltro, il decreto legislativo prevede come strumenti di omogeneizzazione di queste normative la concertazione con gli organismi di rappresentanza datoriale e sindacale, nonché il parere

avanziamo proposte molto innovative, che attengono, di nuovo, alle pari opportunità tra uomini e donne: proponiamo di introdurre un congedo paterno obbligatorio quando nasce un figlio e di modificare la legge sui congedi parentali in maniera da renderli più convenienti e meno penalizzanti anche per i padri, per gli uomini che vogliono andare in congedo, in un periodo di tre anni, per prendersi cura del figlio. del figlio. Questo è uno dei grandi problemi che riguardano le pari opportunità, perché sappiamo tutti che tra i maggiori handicap per l'entrata delle donne nel mercato del lavoro e per la loro permanenza nell'ambito delle carriere e delle professioni vi sono proprio la maternità e la cura. C'è un dato drammatico, che parla di una donna su cinque che è costretta a lasciare il lavoro quando nasce il primo figlio, e questo per la scarsità, spesso per la mancanza totale di servizi, e perché il lavoro di cura grava quasi tutto sulle spalle delle donne. Anche in proposito abbiamo dati che vorrei rendere noti a chi non li conoscesse: le donne dedicano alla cura 5 ore e 20 minuti al giorno in più rispetto al lavoro fuori casa, gli uomini, quando va bene, un'ora e 35 minuti. Il disequilibrio è davvero troppo e insopportabile. Vorrei anche comunicare un fatto di nuova cultura, che riguarda il lessico, se volete: ma qui, davvero, il lessico è sostanza. Parliamo di conciliazione fra maternità, lavoro e carriera, e di condivisione. La condivisione per noi è il vero traguardo su cui lavorare per liberare il tempo per la donna e realizzare quindi uno scambio tra un maggiore spazio pubblico per la donna e un maggiore spazio da dedicare alla cura per l'uomo: occuparsi di un figlio, di un bambino come fanno le mamme sarebbe davvero un grandissimo arricchimento anche per gli uomini. Mi ha sorpresa molto positivamente la recente sentenza del tribunale di Firenze che ha riconosciuto ad un padre la possibilità di andare in congedo anche nei due mesi che precedevano il parto della moglie, e questo per occuparsi del nascituro, e non soltanto della salute della madre. Quindi, conciliazione e condivisione: questo davvero è il nuovo traguardo per una donna moderna in una famiglia moderna. È il nostro orizzonte culturale e vorremmo che non fosse un'utopia. Per quanto riguarda i congedi parentali, sappiamo che solo il 6 per cento dei padri ne fruisce, sia per ragioni culturali (a volte gli uomini che vanno in congedo parentale vengono derisi dei colleghi: questa è realtà, è storia) sia perché non è economicamente conveniente, perché in genere all'interno della coppia è l'uomo che guadagna di più, ed avere una riduzione dello stipendio al 30 per cento è penalizzante per quella coppia e quella famiglia.

non dover scegliere tra lavoro, carriera e maternità e che vogliono davvero avere eguali opportunità lungo tutto l'arco della vita. Per questo invito l'Assemblea, e possibilmente anche qualche collega della maggioranza, a votare favorevolmente su questi emendamenti.

esperienza diretta) da parte dei sindaci delle più varie forze politiche e che governano giunte dei più diversi colori politici

dall'articolo 54 del Testo unico degli enti locali e dal suo troppo vasto regolamento, quello cioè che fa riferimento alla sicurezza urbana. Si emanano ormai ordinanze sui temi più disparati

singolari provvedimenti ed ordinanze di deislamizzazione di piccoli Comuni montani. Il tutto per dire, signor Presidente, che credo che il Ministro dell'interno debba un po' riflettere su tale questione e verificare l'uso del potere di ordinanza, così come definito nell'ultimo testo di sicurezza urbana, affinché i sindaci in nessun modo

mentre noi qui dentro dibattiamo, fuori da quest'Aula ci sono lavoratori precari

Roma, titola: «La protesta dei precari dell'ISPRA: a rischio cinquecento posti». Voglio ricordare che l'ISPRA è l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale che da ieri mattina alcuni di questi ricercatori sono sul tetto dell'ente. Cosa chiedono? Lottano contro il precariato non scenderanno finché non avranno certezze sul futuro e la stabilizzazione del contratto. Voglio ricordare che l'ISPRA a Roma ha tre sedi e 1.000 dipendenti; a giugno ha mandato a casa 250 precari e per altri 250 per altri 250 dovrebbero arrivare lettere di licenziamento. Insomma, il 40 per cento del personale, la quasi totalità dei lavoratori giovani dell'ente, non potrà più svolgere il lavoro che porta avanti da anni. Rischiano così di saltare importanti progetti come il MOSE di Venezia e di finire chiuse in un cassetto le ricerche sulle biodiversità marine o sul monitoraggio ambientale nelle aree di scarico delle piattaforme industriali e sulla cosiddetta nave dei veleni in Calabria. Signor Presidente, comprendo che qui dentro noi dibattiamo e magari votiamo seguendo gli ordini di scuderia, ma uno sforzo in più per la ricerca, per trovare i fondi, per alleviare le sofferenze di questi lavoratori bisogna farlo. Lo ricordo ancora una volta: questa è un crisi lunga e difficile.

questi lavoratori non possono essere lasciati soli, non devono essere abbandonati. Noi siamo con loro e auspico che anche la maggioranza possa fare di più per salvaguardare le giuste istanze di chi protesta per il posto di lavoro e per un tozzo di pane. **Sugli Presidente, vorrei sollevare il problema del funzionamento delle Commissioni, in particolare delle Commissioni bicamerali.

dedicano anche un'ora o due del loro tempo a cercare di immortalare i senatori in posizioni strane che possono essere assunte

Io credo che la Presidenza e i colleghi dovrebbero riflettere su questa prassi che, francamente, alle volte mi fa pensare di essere quasi un animale in gabbia fotografato da professionisti che, per carità, fanno il loro lavoro, ma che finiscono per rendere ridicola un'istituzione importante per la vita democratica del nostro Paese. Chiedo alla

anche della maggioranza. In particolare, il nostro Gruppo ha presentato un'interrogazione sulla grave vertenza e sulla situazione che si sta creando con riferimento ai cantieri navali di Castellammare una delle zone che ha fornito e fornisce tuttora le migliori produzioni cantieristiche del nostro Paese. In seguito ad una crisi aziendale

per affrontare i temi relativi al recupero del tessuto produttivo di una realtà storicamente oltre che quantitativamente e socialmente rilevante. Nel frattempo il il Governo ha già delineato un percorso per creare un clima tale da consentire che la vicenda possa essere affrontata con maggiore tranquillità e serenità da parte dei lavoratori. Ieri abbiamo sottoscritto con la Regione Campania

di circa 1.800 lavoratori (se non di più) altrimenti privi di strumenti di garanzia e di tutela. Questo al fine di costruire un clima che consenta, in sede di Ministero dello sviluppo economico, ma non solo, di affrontare con minore pressione